Comunico che in data 18 gennaio 2024 è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro delle imprese e del* made in Italy*, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali* «Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico»

provvedimento importante che ha animato la discussione prima in Commissione e dopo in quest'Aula. Chi ha seguito i lavori dell'Assemblea sa che siamo probabilmente all'atto conclusivo di un teatro dell'assurdo, cui si è abbandonato il senso del razionale e si è rifiutato un linguaggio logico-consequenziale, perché la comunicazione politica sovverte il principio della realtà, dimenticando che il principio dell'autonomia è previsto nella nostra Costituzione e che la funzione di programmazione e coordinamento da parte dello Stato è un principio ordinatore della funzione, non un freno alla libertà delle articolazioni territoriali. Il Gruppo Azione ha sempre cercato di interpretare un'opposizione nel merito delle cose. Siamo fieramente all'opposizione di questo Governo, ma se una cosa è giusta, anche se viene fatta da un Governo al quale siamo in opposizione, noi non ci tiriamo mai indietro. Se possiamo fare qualcosa di positivo per l'Italia per migliorare un provvedimento noi ci siamo e lo abbiamo dimostrato in diverse occasioni. diverse occasioni. Dicevo che è un teatro dell'assurdo perché, dopo questo voto, ci sarà chi dirà che finalmente, dopo anni, è stata realizzata l'autonomia,

perché questa riforma spaccherà in due l'Italia, come non fosse già divisa da divari territoriali sempre più difficili da colmare e sempre più insostenibili, le riforme del PNRR non dovessero servire in primo luogo per ridurre le disuguaglianze tra il Sud e il Nord, tra il centro e le periferie. Ecco, entrambe le posizioni per noi sono ideologiche e per questo sbagliate. Innanzitutto dobbiamo dire che questa legge quadro, che farà entrare in vigore il tema dell'autonomia differenziata, diventerà realtà se e quando saranno finanziati adeguatamente i livelli essenziali di prestazione. In secondo luogo, In secondo luogo, proprio per riportare il dibattito a un principio di realtà, è giusto ricordare che il processo di autonomia era stato già avviato, per esempio, dal Governo Gentiloni nel febbraio 2018, in una versione che conteneva disposizioni per il Mezzogiorno non molto dissimili da quelle qui contenute oggi e migliorate per il lavoro svolto, anche dalle opposizioni, in sede di Commissioni. Dunque, con la serietà e la responsabilità verso il Paese che da sempre ci animano, nell'interesse del nostro dibattito, noi non ci presteremo a questo gioco delle parti. Noi non siamo qui per dire che l'autonomia è un male e sapete perché? Perché non lo è, perché è prevista dalla nostra Costituzione. Noi siamo qui per dire che delegare alcune funzioni alle Regioni è giusto e che ha un senso, perché l'autonomia può essere un'opportunità di crescita anche per il Sud. Dipende dalla capacità di governare, dipende dalla fame di riscatto, dipende dalla voglia di correre, come ci ricorda un giurista illuminato come Sabino Cassese. quindi pensare che il tema dell'autonomia differenziata possa essere un vessillo solo per le Regioni del Centro-Nord. Ciononostante, la proposta di questo Governo non ci convince pienamente. Dove sono i Senza troppi giri di parole, avreste dovuto dirci chiaramente quali intendevate finanziare e come. Nel testo si prevede un termine di ventiquattro mesi, ma ad oggi, per i LEP, questo Governo non ha previsto un euro. Questo è corretto, per riportare il dibattito al principio di realtà. Noi sosteniamo che prima debbano essere finanziati adeguatamente i LEP e che dopo debba entrare in vigore il tema dell'autonomia differenziata. Il Governo Meloni avrebbe potuto proseguire in questo senso, nella strada già istruita dal Governo Draghi, che aveva finanziato un LEP, quello relativo agli asili nido, e che in qualche modo aveva indicato una strada che era corretta da seguire per dare concretezza al tema dell'autonomia differenziata.

Votare oggi a favore del provvedimento significherebbe firmare una delega in bianco e noi, mi dispiace, ma non ci fidiamo delle buone intenzioni o delle vostre intenzioni. Noi ci fidiamo dei fatti. Noi ci fidiamo delle azioni concrete. Perché non votiamo contro? Perché noi non crediamo Perché noi non crediamo che il principio dell'autonomia sia una strada divisiva per l'Italia. Se tale principio fosse stato fatto in maniera seria, in maniera ordinata,

di colmare i divari tra le Regioni del Sud e le Regioni del Nord, tra il centro e le periferie. Per questo motivo, dichiaro il voto di astensione da parte di Azione al provvedimento sull'autonomia differenziata.

Presidente, colleghi, oggi ci apprestiamo a votare il disegno di legge sull'autonomia differenziata. Stiamo vivendo una giornata, per quello che mi riguarda, storica. Lo dico da veneto, lo ammetto, anche con un po' di emozione. Con questo voto di oggi, con il centrodestra al Governo, Governo, realizziamo la volontà dei cittadini: penso in modo particolare ai 2,3 milioni di veneti e ai 2,9 milioni di lombardi che hanno votato, in occasione del *referendum*, a favore di questa riforma. una riforma che dunque è un risultato e, oserei dire, una grande vittoria dei cittadini per i cittadini. Non è un caso che siano 14 le Regioni che, a diverso titolo, hanno chiesto maggiore autonomia allo Stato, deliberando di avviare una trattativa col Governo centrale. Riformare e modernizzare le nostre istituzioni: oggi, con questo voto, realizziamo appunto la volontà dei cittadini. Ecco perché questo è un passaggio storico ed epocale, nella storia

Al contrario, l'opposizione - posizione che chiaramente rispettiamo - anziché guardare al futuro, preferisce lasciare tutto così com'è, optando per l'immobilismo e la conservazione. L'autonomia è nella storia dell'Italia. Un grande Padre costituente, che fu anche Presidente della Repubblica, Luigi Einaudi, disse che si sarebbe dovuto garantire a ogni uomo l'autonomia che gli spetta e, quindi, a ogni territorio. Un altro protagonista della nostra storia, il siciliano don Luigi Sturzo, affermò: «sono unitario, ma federalista impenitente». Einaudi e don Sturzo, due figure centrali nella storia repubblicana, ci dicono quanto siano profonde le radici dell'autonomia. Sono le radici di una riforma culturale, che oggi impone un cambio di mentalità. L'autonomia è un impegno, è un primo passo concreto, che va finalmente nella giusta direzione. Ricordo che il regionalismo differenziato si pone in continuità e in sintonia con le caratteristiche territoriali della nostra Italia, Italia, che è un mosaico di territori, dalle potenzialità straordinarie. Le esigenze delle Regioni sono diverse e ciascuna di esse, grazie al disegno di legge in esame, potrà ottenere e gestire alcune materie, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi nei confronti dei cittadini. L'autonomia è responsabilità: la conseguenza più importante di questa riforma è riassunta in questa bellissima e semplicissima parola, «responsabilità». In parole povere, il cittadino ha il diritto di sapere chi gestisce la cosa pubblica come lo fa, in modo che sia egli stesso a giudicare chi amministra bene e chi amministra male, senza inutili e normali scaricabarile. È un concetto che è stato anche ben evidenziato dall'autorevole costituzionalista Sabino Cassese, che presiede il comitato per i LEP, che ha svolto un importante e proficuo lavoro per la loro determinazione, che non era mai stato fatto prima d'ora.

Fra le disposizioni assunte all'unanimità - lo sottolineo: con il voto di tutti i partiti - c'era la necessità di procedere a una legge quadro, che coinvolgesse il Parlamento; inoltre, si è stabilito che si sarebbe dovuti arrivare alla definizione dei LEP

era lo *step* necessario, come ha detto il professor Cassese; per finanziare qualcosa, occorre prima definire quello che si vuole finanziare e stabilirne il livello essenziale, e noi lo abbiamo fatto.

Noi vorremmo stabilire un principio: la pubblica amministrazione sia più vicina possibile ai bisogni e alle esigenze dei cittadini, al principio di sussidiarietà. Vogliamo che l'autonomia differenziata avvenga con le giuste e dovute garanzie, con il contributo del Parlamento, assicurando l'uniformità dei diritti essenziali a tutti i cittadini, da Nord a Sud. È qualcosa di rivoluzionario e sapete perché? Perché questa riforma individua un corretto bilanciamento tra il principio di autonomia finanziaria e quello di solidarietà con il sistema perequativo e il suo funzionamento. Perequazione e solidarietà in questo provvedimento ci sono. Nel dibattito sull'autonomia, più volte si è detto che il Parlamento avrebbe assunto un ruolo di spettatore passivo. Non è così e lo dimostra il fatto che la determinazione dei LEP sarà affidata a norme di rango primario, che devono quindi passare all'esame delle Camere. Lo dimostra il fatto che la legge di approvazione delle intese è rafforzata, ovvero deve avvenire a maggioranza assoluta dei propri componenti. Oggi viviamo nel XXI secolo e il ruolo dello Stato e delle Regioni è cambiato in questo primo quarto di secolo rispetto al passato. Com'è cambiato? Com'è cambiato? Penso ad esempio all'emergenza Covid, alla collaborazione che c'è stata tra Stato e Regioni, e credo che votando quest'autonomia abbiamo l'intenzione di guardare al futuro. Colleghi, non possiamo guardare al futuro con lo specchietto retrovisore: ecco perché oggi bisogna lavorare a un nuovo modello di coordinamento tra politiche statali e regionali, con l'obiettivo di rendere più efficiente il raccordo tra Stato e Regioni. Mi avvio quindi alle conclusioni. Con questo Governo e con questa maggioranza in Parlamento abbiamo deciso di non rimandare alle calende greche la volontà espressa dai nostri cittadini. In maniera coesa e compatta abbiamo mantenuto un impegno assunto con gli italiani. L'autonomia non è un capriccio: non è un caso, come dicevo prima, che 14 Regioni ordinarie su 15 chiedano l'autonomia; non è un caso che lo abbiano chiesto anche governatori di centrosinistra, che hanno solo un interesse prioritario: dare maggiori servizi alle proprie comunità. Da oggi comincia un percorso nuovo di rinascita delle nostre istituzioni. Diciamo sì a una riforma che premia chi amministra bene e quindi vuol dire prima di tutto responsabilità. Diciamo sì a una riforma che guarda al bene e al futuro delle nostre comunità e che serve soprattutto per dare più

un'autonomia che è diventata un modello non solo per aver sanato le ferite della storia - ricordo che siamo una minoranza linguistica passata allo Stato italiano a seguito della Prima guerra mondiale - ma anche per aver saputo garantire benessere economico e sociale alla nostra terra. Ricordo che l'Alto Adige, dopo le due guerre mondiali, era una delle terre più povere in Europa e grazie all'autonomia è stata portata in poco tempo ai più alti livelli del nostro Continente. Tanti sono coloro che individuano nell'autonomia altoatesina un esempio virtuoso, un modello di pace da applicare anche in ambito internazionale per la risoluzione di conflitti etnici. Se guardiamo a quello che accade in Israele o in Ucraina, scopriamo il valore di quanto è stato costruito in tutti questi anni. Ma cosa significa autonomia? Autonomia significa innanzitutto scelte politiche più vicine ai cittadini; è la riduzione della distanza tra i cittadini e i luoghi della decisione; è la possibilità di costruire politiche in linea coi bisogni del territorio e decisioni migliori e più adeguate alle esigenze locali. Autonomia significa però anche assunzione di responsabilità e garanzia di efficienza; vuol dire rispondere delle proprie scelte senza potersi appellare o poter dare la colpa allo Stato centrale; implica una maggiore responsabilità che investe le pubbliche amministrazioni e anche i cittadini rispetto alle scelta della propria classe dirigente. L'autonomia è quindi soprattutto un abito mentale diverso da quello attuale e richiede un cambio di prospettiva. Condividiamo questi principi, signor Presidente, perché il nostro partito ha sempre guardato con grande interesse a tutte le varie riforme in chiave federalista portate avanti in questi anni. Lo abbiamo fatto perché pensiamo che questo impianto convenga ad un Paese come l'Italia, che nelle forti identità di ogni Regione ha il suo punto di forza. Il testo che oggi stiamo per votare non è una modifica costituzionale, ma l'attuazione della riforma del 2001. Ci sono voluti ben ventitré anni per dare seguito a un precetto costituzionale. Questo tempo così lungo ci ha permesso di maturare un giudizio completo su quella riforma del Titolo V, che, con le materie concorrenti, ha portato un incremento importante dei contenziosi tra Stato e Regioni a statuto ordinario davanti alla Corte costituzionale, per la natura stessa delle materie concorrenti, i cui confini non sono mai stati di semplice definizione. Il problema non ha riguardato solo le Regioni a statuto ordinario, ma anche le autonomie speciali. Da questo punto di vista, il caso dell'Alto Adige è paradigmatico: in seguito alla riforma costituzionale del 2001, per via di una serie di sentenze della Corte costituzionale, i suoi *standard* di autonomia si sono drasticamente ridotti, tanto da essere ben lontani da quelli del 1992, sulla cui base l'Austria rilasciò la quietanza liberatoria all'ONU per dichiarare chiusa la questione sudtirolese.

Non condivido infine le critiche di coloro che vedono in pericolo l'unità e la stabilità del Paese, in primo luogo perché l'articolo 5 della Costituzione, che rappresenta uno dei pilastri fondamentali del nostro ordinamento, sancisce il principio che la Repubblica è una e indivisibile. Inoltre, la potestà legislativa esercitata dalle Regioni ai sensi dell'articolo 117 trova il limite invalicabile del rispetto della Costituzione. Anche le intese di cui al presente disegno di legge sono sottoposte, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, all'approvazione delle Camere a maggioranza assoluta. Rimane poi comunque pur sempre il limite minimo dei LEP. Su questo ha ragione la collega Gelmini, quando dice che quello dei LEP non è più un discorso aggirabile: è una fatica che si sarebbe dovuta fare in questi vent'anni e non perché sia legata al regionalismo differenziato, ma perché la loro determinazione è questione generale di tutela dei diritti civili e sociali di tutto il Paese. Il presente disegno di legge non è quindi la fine del mondo; al contrario, riteniamo che sia un importante passo in avanti, che richiede però ancora tanto lavoro affinché le intese diventino possibili e in grado di migliorare la qualità complessiva della vita dei cittadini. Noi, come SVP, per la nostra storia e cultura politica, non possiamo che esprimere un voto favorevole.

il disegno di legge recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario che ci accingiamo a votare è un provvedimento che nasce da lontano e certamente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 Costituzione ha poi trovato una sua esplicazione nella successiva riforma del Titolo V della Costituzione che, come sappiamo, ha modificato l'articolo 116, aprendo la strada all'autonomia delle Regioni che sono state poi ripartite in un'autonomia esclusiva, un'autonomia concorrente o ripartita e una capacità di legiferare semplicemente in attuazione delle leggi dello Stato. Con questa premessa, voglio dire che certamente condividiamo pienamente con il ministro Calderoli che questo provvedimento ha origini lontane e trova una piena legittimazione costituzionale nella misura in cui in esso si dichiara di voler dare attuazione all'autonomia delle Regioni nelle materie in cui è già stata loro riconosciuta potestà legislativa esclusiva, e fin qui siamo d'accordo. Tuttavia, premesso e chiarito che l'impianto normativo di questa legge e le sue finalità astratte sono pienamente legittimi e condivisibili, le modalità con le quali questo Governo ha inteso dare attuazione all'autonomia differenziata per le Regioni a Statuto ordinario non ci convincono. Non ci convincono perché risultano divisive e sperequative e perché causeranno la frammentazione del territorio nazionale in tante Regioni, ognuna delle quali potrà avere regole diverse, per esempio in materia di istruzione, trasporti, sanità, edilizia o risorse energetiche, soltanto per citare gli argomenti più importanti. importanti. Sgombriamo subito il campo allora da un equivoco: la finalità autonomista è legittima e condivisa, ma la sua attuazione, così com'è stata concepita, non va bene, perché - mi dispiace dirlo - prende un'accezione separatista e si traduce in sostanza nella negazione del principio di solidarietà economica e sociale che costituisce uno dei capisaldi della nostra Repubblica. Non si illudano le Regioni del Nord, pensando che questa legge finalmente darà loro pieni e liberi poteri di esercitare la spesa, perché quest'apparente autonomia che verrà riconosciuta con la sottoscrizione delle intese avrà un prezzo molto alto, che è fissato nell'articolo 8 del testo che ci accingiamo a votare, in cui viene sancito che dall'applicazione della presente legge e di ciascuna intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In parole semplici, questo significa che le risorse economiche per attuare l'autonomia delle Regioni non ci sono. Devono essere le stesse Regioni che vogliono sottoscrivere le intese a individuare le risorse per garantire i LEP nelle materie per le quali hanno richiesto l'autonomia differenziata: come si attuerà quindi quest'autonomia? Con il gettito di uno o più tributi locali che verranno trattenuti nei territori e utilizzati per garantire i LEP, i famosi livelli essenziali delle prestazioni. dunque che le Regioni che hanno un tessuto economico e sociale più avanzato e producono un maggior gettito tributario avranno maggiori possibilità di garantire questi LEP utilizzando i propri tributi, mentre quelle con un'economia arretrata, dove l'economia locale non ha grandi gruppi industriali o insediamenti produttivi e il gettito tributario è composto dalle imposte pagate dalle famiglie e dalle piccole imprese, avranno a disposizione risorse ridotte per garantire i LEP. Già così mi sembra evidente che questa legge sia fatta male, sia fatta male, ma non basta: i livelli essenziali delle prestazioni, che riguardano i diritti civili e sociali, non sono stati ancora determinati, per cui non è dato neppure sapere quale sia effettivamente il loro costo. La legge che stiamo discutendo adesso prevede espressamente che prima di poter riconoscere l'autonomia differenziata alle Regioni che ne faranno richiesta sarà necessario determinare i LEP. Giustissimo,

La prima è che senza la determinazione dei LEP le Regioni che vogliono l'autonomia differenziata non potranno neppure avanzarne richiesta e dovranno aspettare che la Commissione proceda alla loro determinazione e quantificazione, quindi ritorniamo a quello che ci siamo detti anche in sede di discussione generale: quale urgenza c'era di portare questo provvedimento così insistentemente in Parlamento, se ancora non sappiamo qual è il valore dei LEP? La seconda ragione è un piccolo intralcio che nel testo normativo è entrato a seguito dell'intervento delle opposizioni nel corso della discussione generale in Commissione,

è evidente che questo enunciato - ossia che dovranno essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale - finisce per avere un valore un valore programmatico: si limita cioè a dire che i LEP devono essere garantiti ugualmente su tutto il territorio nazionale, ma si scontra evidentemente con un altro enunciato collocato nell'ultima parte della legge, che invece stabilisce che dalle attuazioni delle disposizioni di questa legge non devono derivare maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica. Mi sembra che siamo in un cortocircuito narrativo, istituzionale e delle disposizioni. Questo cortocircuito è talmente evidente che lei stesso, signor Ministro, alla fine ha assicurato, con pubbliche dichiarazioni, che i LEP verranno finanziati e che verranno trovate le risorse per garantire effettivamente che i diritti civili e sociali di cui essi costituiscono espressione siano garantiti equamente. Peccato però che in questa legge non si ravvisi una sola norma in cui si indichi la fonte per garantire questa risorsa economica. In quest'Aula ho più volte sentito dire, soprattutto dai colleghi della maggioranza, che quello in esame è un disegno di legge procedurale, cioè servirebbe soltanto a definire le procedure con le quali le Regioni a statuto ordinario potranno chiedere il riconoscimento dell'autonomia differenziata. Mi dispiace osservare però che non è così: questo non è un disegno di legge procedurale. Certamente nelle intenzioni iniziali del Governo era così, si sarebbe dovuto trattare di una legge procedurale, tanto che il testo originario prevedeva l'invarianza di spesa e che le risorse per attuare l'autonomia differenziata fossero tutte a carico delle Regioni richiedenti. Molto facile, in teoria, ma poi in Commissione si è visto che così semplice non era e non lo era neanche per i partiti della maggioranza, non per tutti loro. Il testo modificato grazie a un intenso lavoro

e, come tutte le leggi, deve avere le sue risorse, che in questo caso invece mancano, anzi addirittura sono escluse. Ho sentito dire in quest'Aula, ripetendo un *refrain* che va avanti da anni, che è giunta l'ora che le risorse vengano date a chi è capace di spenderle. Anche qui però, signor Ministro, questo Governo fin dal suo insediamento ha sistematicamente sottratto le risorse al Sud. Partiamo dal fondo di perequazione, ridotto da 4,4 miliardi a 800 milioni di euro. Pensiamo alla rimodulazione del PNRR, con 10 miliardi sottratti ai Comuni, soprattutto delle isole. Parliamo anche di 1,6 miliardi che dal Fondo sociale di sviluppo e coesione sono stati depredati alla Sicilia e alla Calabria, per essere portati sul Ponte sullo Stretto. Sono saltati anche i finanziamenti destinati al contrasto del dissesto idrogeologico e alla realizzazione dell'autostrada Siracusa-Gela. Insomma, questo Governo ha sottratto risorse al Sud per un valore equivalente a circa 15 miliardi di euro. Come vogliamo pensare di realizzare un'autonomia differenziata, quando si sottraggono sistematicamente le risorse al Sud, le si destinano al Nord e poi si dice ognuno faccia da sé? Non funziona così. Le conclusioni di questo mio intervento, Presidente, le voglio affidare a una vicenda realmente accaduta in tempo di Covid, che mi è venuta in mente proprio ascoltando le repliche del ministro Calderoli la settimana scorsa, in seguito alla discussione generale.

non ci sono posti letto per curarlo, perché tutte le rianimazioni dei vari ospedali sono piene; entra allora in funzione il nostro sistema sanitario nazionale e con un volo militare Ettore Consonni viene trasportato all'Ospedale Civico di Palermo, dove viene ricoverato in rianimazione, curato e salvato. e salvato. Dopo un mese di coma, si sveglia incredulo: si era addormentato a Bergamo, ma si è svegliato a Palermo; all'inizio - lo racconta lui stesso - pensava a uno scherzo del personale sanitario, poi si convince effettivamente di essere finito a Palermo. Dopo un anno ritorna in Sicilia e addirittura,

veneta, con un eccellente servizio pubblico, laddove invece le cure che avrebbe potuto ricevere altrove sarebbero state a pagamento. Questa storia mi viene in mente perché, come lei ha giustamente ricordato, la sanità veneta l'ha curata gratuitamente. Io le chiedo: con la sua autonomia differenziata, cosa sarebbe successo a Ettore Consonni? Se ogni Regione dovrà investire nei LEP...

sindaci, amministratori, comitati, associazioni e sindacati, che anche in questi giorni si sono ritrovate in molte piazze del Paese e assieme alle quali diciamo oggi, in quest'Aula, che non intendiamo fermarci qui. *(Applausi)*. Questa discussione non finisce in Parlamento, dove i numeri, come sappiamo, sono quelli che sono. Noi crediamo che sia nostro dovere politico lavorare tutti, a partire dalle forze di opposizione, naturalmente, per indire un *referendum* abrogativo *(Applausi)* che dia ai cittadini la facoltà di bocciare questa scellerata e sciagurata riforma.

ma più in generale per tutti i cittadini, anche certamente quelli che al Settentrione vivono in una condizione difficile e di sofferenza sociale. Dovevate pagare un prezzo alla Lega, lo state facendo sulla pelle non solo di questo Parlamento, ma dei principi fondamentali della Costituzione repubblicana. Avete fatto uno scambio scellerato tra i partiti della maggioranza: l'autonomia differenziata in cambio del premierato, due riforme apparentemente opposte il massimo del decentramento, da un lato, e il massimo dell'accentramento, dall'altro - che hanno però in comune la definitiva marginalizzazione del Parlamento *(Applausi)*, un'autentica torsione della nostra democrazia. Noi non ve lo consentiremo. Gireremo l'Italia, raccoglieremo le firme che servono per il *referendum* abrogativo, sosterremo i comitati - che oggi ringrazio molto per il lavoro svolto in questi anni - e soprattutto vi chiameremo come meritate. vi ho già detto una volta, vi chiameremo Fratelli di mezza Italia e vi chiameremo Lega Padana. *(Applausi)*. Questo è infatti quello che avete scelto di essere. So bene, Presidente, questo provvedimento è il frutto di una lunga stagione politica, con un salto di qualità però ancora più grave. Rivendico in quest'Aula di aver fatto parte di quella sinistra che giustamente nel 2001 si oppose alla riforma del Titolo V della Costituzione. Considero però molto positivo che in questi mesi sia cresciuta tra le forze di opposizione la consapevolezza di un cambio di rotta, anche alla luce dell'esperienza di questi anni. Cos'è stata la pandemia, se non la drammatica testimonianza che un Paese frammentato non ha gli strumenti giusti per reagire, per esempio, alla più grande delle emergenze? E ancora, come si fa a non vedere che la diseguaglianza è diventata la cifra del nostro tempo, se dove vivo io l'aspettativa di vita è inferiore di quattro anni rispetto a quella nel Nord Italia? Se i diritti non sono gli stessi per tutti, allora vuol dire che questa strada porta verso un burrone. È per questo che nei mesi scorsi abbiamo sostenuto, firmandolo, il disegno di legge popolare di riforma degli articoli 116 e 117 della Costituzione, che quest'Assemblea colpevolmente ha scelto di esaminare solo dopo la riforma del Governo, perdendo un'altra gigantesca occasione. Noi non siamo contro il regionalismo, Presidente, ma lo immaginiamo - come nell'articolo 5 della Costituzione - in stretta connessione con i principi contenuti nella prima parte della Carta: un regionalismo solidale, il contrario, cioè, di questo impianto egoista, competitivo e secessionista che è alla base della vostra riforma *(Applausi)*, un progetto devastante per il Sud, ma anche per il Nord. Davvero pensate che un'Italia divisa in venti piccoli Stati, che vivranno l'uno contro l'altro, possa essere la risposta giusta alle sfide del mondo di oggi? Un'Italia con differenti diritti, con le gabbie salariali e con sistemi amministrativi diversi? Davvero pensate che un cittadino che oggi per curarsi deve andare dal Sud al Nord, perché il suo diritto alla salute non è uguale dappertutto, vedrà migliorata questa sua condizione con l'autonomia differenziata? Non vi viene il dubbio che in questo modo le Regioni povere diventeranno ancora più povere? I divari cresceranno ancora, inevitabilmente, e non sarà certamente la foglia di fico dei cosiddetti livelli essenziali delle prestazioni a sanare la situazione. Ve l'ho già detto più volte in quest'Aula: i livelli delle prestazioni dovrebbero essere uniformi più che essenziali *(Applausi)*, come c'è scritto nel disegno di legge di iniziativa popolare. Soprattutto, non è sufficiente definire i LEP, se poi si dice che la spesa pubblica deve rimanere invariata. Non ha alcun senso parlare di livelli essenziali delle prestazioni se non ci dite come saranno finanziati *(Applausi)*, quando tutti sappiamo, peraltro, che per ridurre i divari servirebbero risorse assai importanti, che non ci sono (o, meglio, che non si vogliono trovare). Continuate infatti a portare avanti sempre le solite ricette liberiste, come avete fatto negli anni e nei decenni passati. una foglia di fico, insomma, che conferma la storia di questi anni, perché un equivalente dei LEP in materia sanitaria esiste già: sono i livelli essenziali di assistenza, già definiti da anni, ma comunque inefficaci, perché non sufficientemente finanziati.

per poi dare rassicurazioni, ma solo a parole, che la scuola non sarà frammentata. Mi dispiace, Ministro, gliel'ho già detto: non ci bastano queste rassicurazioni, non ci bastano queste parole. Consideriamo grave, gravissimo che si possa anche soltanto immaginare un percorso formativo diverso, più o meno inclusivo, a seconda di dove si ha la fortuna di nascere. Noi crediamo che debba essere salvaguardato il carattere unitario e nazionale del nostro sistema pubblico d'istruzione, che è un fondamento sul quale si costituisce e si dovrebbe costituire la cittadinanza. La scuola della Repubblica in questi anni è stata già troppe volte colpita da riforme sbagliate; non datele il colpo di grazia finale, Ministro, perché non riguarda semplicemente il presente, ma il futuro di questo Paese e delle sue generazioni più giovani.

Signor Presidente, voglio partire da un punto cruciale. Qui in Forza Italia abbiamo un credo: libertà individuale, principio di sussidiarietà Stato meno ingombrante, ma c'è un "ma"; questo disegno di legge sull'autonomia ci ha fatto riflettere, è un tema che tocca le corde del cuore, soprattutto per chi come me è del Sud. In verità, non sarebbe cambiato nulla, neanche se fossi stato un parlamentare del Nord, per rispetto dei principi di solidarietà nazionale ed equità sociale che devono riguardare tutti i cittadini italiani. Non possiamo ignorare però che ogni decisione che riguarda l'autonomia implichi anche una riflessione sul Sud dell'Italia e sulla questione meridionale. Non c'è uno sviluppo autentico del nostro Paese, se una parte rimane indietro.

cioè le mettiamo una cornice, come dice il senatore Romeo, valorizzandone i contenuti e collegandola strettamente ai diritti di cittadinanza e ai servizi essenziali. La differenza fondamentale è proprio questa. Abbiamo insistito molto - anzi, lo abbiamo preteso - affinché l'autonomia fosse correlata ai diritti di cittadinanza, garantendo i servizi essenziali, in modo che non dipendano più dalla spesa storica, ma dai fabbisogni *standard* delle popolazioni. Parliamo del diritto alla salute, alla casa, alla scuola, al lavoro e al tempo libero, nonché di spostarsi liberamente. Parliamo anche dei diritti che riguardano il nostro futuro e quello dei nostri figli, la sostenibilità, l'ambiente e la bellezza, che creano nel tempo ricchezza nei territori e sono i pilastri della nostra società. Pensando alla mia esperienza di sindaco e di architetto, dato sempre interessato dei temi che riguardano la città e i diritti dei cittadini, vedo anche un'altra realtà, signor Presidente. Lo Stato ha già delegato la maggior parte di questi servizi essenziali, circa l'85 per cento del costo totale, nel corso dei decenni passati, agli enti territoriali: il trasporto pubblico locale, i servizi sociali, socioeducativi e sanitari, la manutenzione delle scuole, le reti idriche e il ciclo dei rifiuti. Questo è avvenuto senza che fossero definiti i LEP e con finanziamenti trasferiti sulla base della spesa storica, non dei fabbisogni *standard*. Ad esempio, a Cosenza, avevamo dieci asili nido

Chiedo, allora: come può il Sud e come può l'Italia trarre vantaggio da questa riforma? Io sono convinto che l'attuazione del regionalismo differenziato sia utile al Paese nella misura in cui si definisca un punto di equilibrio tra il rafforzamento delle autonomie territoriali e la coesione economica e sociale dei territori, con la garanzia, appunto, del finanziamento dei LEP in ogni Regione.

Dopo aver ascoltato tanti esperti e dopo un lungo confronto, in quella sede sono stati approvati tanti emendamenti, con l'abile guida del presidente Balboni, che ringrazio; ne sono stati

anche nel constatare che un emendamento presentato dall'opposizione, a firma del senatore De Cristofaro, che io avevo ritenuto meritevole

l'orientamento del Gruppo di maggioranza), poi in Aula sia stato votato ed approvato con il voto di tutti, anche di quelli che mi avevano criticato per aver infranto il patto di maggioranza. Chi teme dunque che il Paese possa spaccarsi per questa riforma può dormire tranquillo. Il provvedimento che oggi licenziamo non comporta un allontanamento dal principio di solidarietà nazionale, senatore De Cristofaro. Non potranno essere destinate maggiori risorse ad alcune Regioni a danno di altre per i servizi essenziali,

non solo attraverso la loro puntuale definizione e quantificazione, ma anche con il loro effettivo finanziamento. È qui, accanto a me, il senatore Silvestro, presidente della Commissione bicamerale che si occupa delle autonomie regionali, che ha già avviato un'indagine conoscitiva proprio sui LEP nelle Regioni del Sud. Signor il Paese è già spaccato e il Meridione continua a soffrire proprio a causa di anni di centralismo, fatti di politiche dirigiste e di tagli dei trasferimenti agli enti territoriali. Il centralismo ha prodotto ha prodotto una differenza nelle dotazioni infrastrutturali - meno autostrade, ferrovie ed ospedali - e il dissesto idrogeologico e anche i grandi eventi sono tutti al Nord, mentre al Sud non c'è alcun evento. Adesso ci saranno grandi opere, come il Ponte sullo Stretto e l'alta velocità, che si ferma a Salerno. Il centralismo ha prodotto l'impoverimento della cultura imprenditoriale del Sud, per il ripetersi di politiche assistenzialistiche che hanno contribuito a soffocare l'iniziativa privata, anziché stimolarla a intraprendere progetti d'impresa sostenibili. ha prodotto il fallimento dei poli industriali finanziati dallo Stato, lasciando solo siti inquinati e inquinanti, che devono essere ancora bonificati, dopo decine di anni. In tema di diritto alla salute, si può notare come molti ospedali periferici siano stati chiusi e il personale medico sia oggi molto più ridotto e insufficiente, per i tagli lineari dello Stato centrale Un esempio di cattiva gestione centralistica della sanità è evidente in Calabria, in cui il commissariamento dello Stato per decine di anni non ha fatto che aggravare la situazione. Oggi si sta cercando di porvi rimedio, attraverso un'amministrazione più determinata e incisiva, più vicina

al reclutamento di medici cubani, che hanno salvato la vita di decine di cittadini calabresi, compresi alcuni medici che lavoravano all'interno degli ospedali. Signor Presidente, la mia esperienza di sindaco mi dice che il problema principale del Sud Italia è la mancanza di opportunità di lavoro. I giovani vanno via perché non trovano un'occupazione dignitosa, non per l'autonomia. Ho trovato persone, intere famiglie, che si sono trasferite nella mia città, o sul mare in Calabria o sulle sue bellissime colline, ed erano pienamente soddisfatte della bellezza dei luoghi, della loro vivibilità e quindi anche dei diritti di cittadinanza. Ho parlato con tanti giovani, che sperano di tornare, ma che non trovano lavoro. Questo è il vero problema: non ci saranno mai risorse sufficienti da destinare a un territorio per promuovere lo sviluppo, se mancheranno il capitale umano, le giovani menti, la capacità di innovare e la creatività. La nostra visione dev'essere allora rivolta al futuro, proponendo di mettere in atto un grande piano per l'occupazione giovanile, non con gli strumenti dell'assistenzialismo, ma legandolo alla transizione ambientale e digitale e alle nuove professioni legate all'intelligenza artificiale. Guardando al futuro, possiamo ispirarci al glorioso passato delle nostre città del Rinascimento, in cui autonomia significava fioritura culturale, economica e sociale, una forte coesione sociale e la diffusione di idee umanistiche, un *humus* che ha stimolato la nascita di grandi artisti come Leonardo e Michelangelo e il sorgere del mecenatismo, plasmando definitivamente l'identità della nostra Nazione. In quest'ottica, l'autonomia differenziata non è una rinuncia, né un allontanamento dal principio di solidarietà nazionale, ma la costruzione di un abito su misura, per rispondere meglio ai bisogni dei cittadini nei territori e anche per l'impegno rinnovato di un Paese che deve crescere unito, seppur nelle diversità

al Governo. Con maggiore autonomia, immaginiamo un'Italia ancor più straordinaria, in cui ogni Regione, proprio come le città del Rinascimento, possa esprimere al meglio il suo potenziale. alla Calabria, in cui proprio qualche giorno fa uno scienziato, Georg Gottlob, che si è trasferito da Oxford all'Università della Calabria, un'università all'avanguardia sui temi digitali e dell'intelligenza artificiale, ha detto che si vive benissimo e che l'università è un polo d'eccellenza in quel campo. La Calabria potrebbe dunque diventare un polo d'eccellenza europeo per l'intelligenza artificiale... ...possono valorizzare il loro patrimonio culturale e archeologico e le energie rinnovabili, per uno sviluppo sostenibile. Concludo con un invito, signor Presidente: guardiamo oltre gli ostacoli, crediamo in un'Italia più autonoma, ma unita, ricca nelle sue diversità, ma coesa nel perseguire il benessere di tutti i cittadini.

non vuol dire suonare a ogni manifestazione pubblica l'Inno di Mameli o istituire il Ministero del *made in Italy* o pensare di fare il blocco navale per impedire che arrivino migranti in Italia. Essere patrioti vuol dire soprattutto difendere sempre e comunque il Paese, l'unità nazionale e la nostra Carta costituzionale. Vorrei partire proprio dalla lunga discussione che abbiamo avuto in questi mesi in Commissione e anche in Aula sulla nostra Carta costituzionale. Sono volate accuse reciproche, anche negli interventi che oggi mi hanno preceduto, su chi voleva e chi non voleva quella riforma del Titolo V della Costituzione votata nel 2001. Certamente non la voleva il MoVimento 5 Stelle, che non c'era, però dico: vi è stata servita su un piatto d'argento l'occasione di rivedere quella riforma,

Avete fatto anche un'altra forzatura, scrivendo il cosiddetto disegno di legge Calderoli, collegato alla manovra di bilancio, quando sappiamo bene che non c'è un euro euro e che vi serviva solo come strumento per silenziare l'opposizione, falcidiare gli emendamenti e accelerare la discussione anche durante la sessione di bilancio.

Tutti i soggetti che abbiamo audito si sono detti contrari a questo disegno di legge, da Bankitalia a Confindustria, dai sindacati alla fondazione Gimbe, dalla Corte dei conti alla Conferenza episcopale italiana e a tutti costituzionalisti. Mi chiedo e vi chiedo allora a cosa serva lavorare mesi e mesi in Commissione, se poi andate avanti per la vostra strada senza raccogliere nessuno dei suggerimenti che vi vengono dati, per non parlare

alla luce dei dati pubblicati dall'Ufficio parlamentare di bilancio, da Bankitalia e dalla Commissione europea, che ci hanno detto: attenzione, se voi permettete alle Regioni di trattenere il gettito fiscale, ci saranno meno risorse a disposizione delle altre Regioni. Volevamo fare audizioni audizioni sull'ambito finanziario e non ci è stato permesso, ma questi mesi di tempo certamente vi sono serviti per fare due cose. serviti per finalizzare il vostro scambio politico, perché di questo si tratta: oggi la Lega pianta la sua bandierina sull'autonomia differenziata; domani Fratelli d'Italia la pianterà sul premierato; dopodomani Forza Italia la pianterà sulla riforma della giustizia, questo è lo scambio politico che c'è stato. questi mesi vi sono serviti anche per fare un'altra cosa indispensabile ad avere oggi i numeri in Aula: far metabolizzare questa riforma ai vostri parlamentari del Sud, che avete convinto con emendamenti aggiunti all'ultimo in Commissione, che sono una vera e propria farsa e che prevedono la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni a equilibrio di bilancio, cosa praticamente impossibile. Personalmente, dico ai parlamentari di maggioranza del Sud che oggi non vorrei stare al loro posto, perché stanno tradendo i loro elettori, ai quali avevano promesso di non realizzare l'autonomia.

ma anche il principio sancito dall'articolo 3 della Costituzione, secondo cui la Repubblica deve rimuovere qualsiasi ostacolo che impedisca il pieno sviluppo della persona umana; voi, invece, quegli ostacoli li state rendendo

Mi riferisco a quello che è successo durante la pandemia, quando in Calabria è morta una bambina di due anni perché non c'era una terapia intensiva infantile, mentre in Veneto ce ne sono tre. A questo mi riferisco! Allora voi evidentemente avete scelto di essere, sì, patrioti, ma di 20 piccole patrie, anzi di 20 nuclei dentro 20 piccole patrie, perché a trarre vantaggio da questa spesa pubblica che si libererà saranno pochissimi, una piccolissima fetta della società. Dovreste invece essere patrioti in Europa, dove avete fatto approvare un patto di stabilità che ci costerà 12 miliardi di euro all'anno di nuove tasse e nuovi tagli. *(Applausi)*. Lì dovete fare i patrioti e non andare contromano. Non è vero che tutta la colpa dei divari è del centralismo, perché la riforma del Titolo V è l'unica forma di regionalismo che abbiamo sperimentato e sappiamo che ha fatto MoVimento 5 Stelle oggi votiamo contro questo progetto scellerato di creare uno Stato arlecchino e, come ha detto qualche giorno fa in Aula il mio collega Roberto Scarpinato, non preoccupatevi perché in quest'Aula a difendere il Paese ci siamo noi, a fianco di quella fetta di Paese

ci siamo noi, a fianco di quella fetta di Paese che invece lotta e vuole l'unità e l'uguaglianza. *(Applausi)*. Voi evidentemente siete troppo impegnati a fermare i treni, a sparare con le pistole alle feste di Capodanno e a fuggire dall'Aula quando parla *(Applausi)*, dando al Paese lo spettacolo imbarazzante di una maggioranza che evidentemente ha deciso di abdicare alla guida del Paese. Noi, invece, combatteremo con tutti gli strumenti che abbiamo per difendere l'unità nazionale: viva l'Italia unita!

dopo tanti anni di dibattito in queste Aule parlamentari, ci saremmo aspettati sicuramente un segno di maggior maturità politica nell'affrontare le questioni relative al federalismo e all'autonomia. Purtroppo, assistiamo ancora alla solita retorica dello spacca Paese (la secessione dei ricchi, l'aumento dei divari), senza invece quel processo di maturazione necessario che ha visto per esempio il nostro partito *in primis* passare magari da posizioni di un federalismo spinto verso quello che Matteo Salvini ha chiamato un federalismo ragionevole, ossia una maggiore autonomia ai territori in un quadro di unità nazionale. *(Applausi)*. Questo è quello che la Lega propone e che oggi è in discussione in quest'Aula, mentre abbiamo sentito solo una serie di processi alle intenzioni di cui capiamo poco la necessità. La classe politica avrebbe dovuto capire, dopo tutti questi anni, che è necessario uscire dalla contrapposizione Nord-Sud, perché «*divide et impera*» è sempre stato l'espediente romano per far sì che il Nord non potesse correre e il Sud non potesse crescere e il potere rimanesse sempre a livello centrale, nelle mani di chi davvero lo detiene in tutte le sue forme.

Sui divari è stato ricordato bene dal ministro Calderoli *in primis* che negli ultimi quarant'anni, senza federalismo e senza autonomia, i divari sono aumentati.

modo, ci sono alcune professioni più qualificate che si insediano al Nord e altre meno qualificate che si insediano al Sud e il *gap* infrastrutturale ed energetico che c'è in questo Paese non può certo essere figlio di un federalismo che non c'è mai stato, perché, come diceva il grande professor Gianfranco Miglio, non è il federalismo a provocare la crisi dello Stato nazionale, ma è la crisi di quest'ultimo che trova una risposta nelle soluzioni federali. È quello che questo Paese non ha mai voluto comprendere. *(Applausi)*.

una serie di passaggi con tutti gli attori principali: con il Parlamento e tutte le associazioni, ci sono passaggi anche abbastanza lunghi per arrivare a una vera attuazione, con l'attribuzione e il perfezionamento delle intese. Altro che mortificazione,

per far vedere che già qualcosa si può assegnare, anche in via sperimentale e facendo alcune valutazioni; l'importante è uscire da questo meccanismo che continuate a mettere in evidenza («spacca Italia», «dividi Italia» o «fermate tutto»). Ma fermate tutto cosa? Mantenere lo *status quo* è la condizione peggiore, che aumenterà sempre di più i divari

Colleghi, posso chiedervi un favore? Quando ha parlato la senatrice Castellone, ho chiesto per favore di non interromperla. Gli stessi che hanno chiesto di non essere interrotti, adesso fanno la stessa cosa: scusate, ma non è corretto nei confronti di chi sta parlando. ROMEO Sì, Presidente, vado avanti nel dire che invece rappresenta un'opportunità per tutti quei territori che si vogliono prendere la responsabilità di gestire competenze nelle quali possono esprimere maggiori potenzialità.

nell'assegnazione delle gare, hanno potuto ricavare le risorse necessarie, di cui hanno beneficiato i cittadini dei Comuni interessati dalle opere, sotto forma di agevolazioni in termini di costo inferiore dell'energia elettrica o di infrastrutture sul territorio? Vale anche per le *royalty* che bisogna pagare sulla produzione degli idrocarburi, che ha visto favorire alcune Regioni del Centro e del Sud, *in primis* la Basilicata. Ricordiamo oggi l'impegno, sempre ai tempi del ministro Calderoli,

immaginate se sulla produzione dell'energia le Regioni avessero competenza esclusiva. Pensate alle fonti rinnovabili (eolico e fotovoltaico), che per ragioni geografiche si trovano in una certa area del Paese

mi avvio alla conclusione cercando di recuperare qualche minuto, visto che sono stato interrotto, facendo presente che, se ci sono Regioni come la Lombardia, il Veneto e il Piemonte, che hanno risparmiato sul costo del personale, non riusciamo a capire perché, in fase di carenza di medici, di infermieri e di personale, queste Regioni, pur avendo i soldi, non possano assumere con un tetto di spesa imposto da uno Stato centrale che, anziché fare gli interessi dei cittadini, li danneggia. *(Applausi)*. Presidente, annunciamo ovviamente il nostro voto favorevole e lo facciamo con calma e con i piedi per terra, sapendo che è l'avvio di un percorso, perché ci sarà ancora il passaggio alla Camera e poi bisognerà cominciare a perfezionare queste intese. Mantenendo quindi i piedi per terra, noi pensiamo che oggi sia un giorno importante. Per questo motivo, voglio ricordare sicuramente chi nelle Regioni

ancora Raffaele Cattaneo e tanti altri che hanno votato quella proposta di *referendum*, che hanno consentito al popolo di esprimersi e che oggi consentono di iniziare un percorso importante. Grazie al Governo. Grazie anche al patto di maggioranza di cui noi andiamo assolutamente fieri. Più poteri al *Premier* significa, dall'altra parte, controbilanciare con più autonomia sul territorio. Viva la Lega! Noi esprimeremo un voto

in varie occasioni di assicurare alla Commissione le condizioni per un confronto approfondito, fondato su adeguati elementi di conoscenza. Devo però anche constatare come questo tentativo su questioni centrali di metodo e di merito abbia avuto la peggio e, alla fine, il disegno di legge che stiamo discutendo, a prima firma del ministro Calderoli, presenti contraddizioni e lacune molto serie, oltre che scelte politiche - a nostro avviso - dannose per l'intero Paese. Partiamo dalle questioni di metodo che inevitabilmente si sono ripercosse sul merito.

«dall'applicazione della presente legge e di ciascuna intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». Perché dunque il collegamento? Una risposta purtroppo non l'abbiamo avuta né dal Governo - il ministro Giorgetti si è negato e alla fine non l'abbiamo potuto audire - né dalla Presidenza del Senato, né è stata convocata sul punto la Giunta per il Regolamento, come pure abbiamo chiesto insieme a tutte le opposizioni. Da tale collegamento, onorevoli colleghi, deriva non solo l'aggiramento del divieto di trattazione durante la sessione di bilancio, ma anche una significativa limitazione del confronto per i tempi, che sono stati contingentati, e per il merito, che è stato circoscritto attraverso un richiamo piuttosto disinvolto all'articolo 81 della Costituzione da parte della Commissione bilancio. Quest'ultima ha dichiarato inammissibili emendamenti che cercavano di affrontare una questione centrale: centrale: subordinare l'eventuale devoluzione di competenze legislative a una o più Regioni alla determinazione e all'effettiva attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che - come prescrive la nostra Costituzione - devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Queste inammissibilità hanno impedito alla Commissione affari costituzionali di discutere e valutare nel merito tali emendamenti e soprattutto hanno impedito che fosse possibile ripresentarli in Aula, accompagnandoli magari da adeguate ipotesi di copertura. Anche se erano emendamenti che - a nostro avviso - non dovevano essere dichiarati inammissibili, perché non comportavano in quanto tali onere alcuno per la finanza pubblica, le decisioni di inammissibilità della Commissione bilancio hanno fatto un po' di chiarezza e hanno confermato ciò che da tempo stiamo dicendo: per attuare i livelli essenziali delle prestazioni in tutto il Paese occorrono nuove risorse e il Governo e la maggioranza che lo sostiene non hanno alcuna intenzione di reperirle. il disegno di legge a prima firma Calderoli è una legge ordinaria, la cui forza vincolante sulle leggi che daranno attuazione alle eventuali intese è quantomeno dubbia. dubbia. Una legge ordinaria - com'è noto - non è solitamente in grado di vincolare una successiva legge ordinaria, qual è appunto quella che recepisce le intese, che peraltro dev'essere approvata a maggioranza qualificata. Non sarebbe stato allora più ragionevole ed efficace definire i presupposti e le modalità per l'attuazione dell'articolo 116 con legge costituzionale, come vi abbiamo proposto e come hanno proposto i cittadini con una legge di iniziativa popolare? E ciò tanto più se si ritiene - come anche diversi esponenti della maggioranza paiono ritenere, insieme alla dottrina pressoché unanime - che l'articolo 116 presenti alcune criticità e sollevi dubbi interpretativi e di coordinamento con le altre disposizioni del Titolo V che sarebbe necessario risolvere. Se anche il ministro Calderoli ritiene che, ad esempio, sarebbe irragionevole attribuire a una o più Regioni la competenza legislativa esclusiva a determinare le norme generali sull'istruzione - aggiungiamo noi, insieme a coloro che abbiamo audito - sarebbe altrettanto irragionevole e controproducente attribuire a una o più Regioni la competenza esclusiva a disciplinare la produzione e la distribuzione nazionale dell'energia o le grandi reti di trasporto e navigazione o il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario o la tutela della sicurezza del lavoro e della salute *(Applausi)*, perché non intervenire subito sull'articolo 116 ed escludere tali eventualità? Pensiamo agli effetti che avrebbe sul nostro sistema produttivo e industriale avere venti o quindici diverse discipline di queste materie. Per quanto riguarda la tutela della salute, pensiamo ai danni che arreca ai cittadini e ai bilanci delle Regioni la crescente mobilità dei pazienti, dovuta all'impoverimento delle strutture pubbliche e alle loro eccessive differenziazioni. Vi abbiamo fatto una proposta molto semplice: correggiamo insieme il Titolo V o almeno formalizziamo una sua interpretazione ragionevole, che, ad esempio, escluda differenziazioni nelle materie in cui prevalgono fondamentali esigenze di uniformità e al contempo chiarisca che, in relazione alle altre, si possono trasferire solo specifiche funzioni e solo sulla base di un procedimento rigoroso di verifica degli effetti.

materie citate nell'articolo 116 possano essere attribuite a una o più Regioni nella loro interezza, in violazione della complessiva architettura costituzionale e dello stesso articolo 116, come abbiamo spiegato nella questione pregiudiziale. Avete inoltre proceduto senza chiarire come verranno determinati e resi esigibili i livelli essenziali delle prestazioni. Il materiale che abbiamo fino ad ora potuto consultare è una fotografia abbastanza sfocata della legislazione esistente, che ad avviso del CLEP potrebbe essere astrattamente considerata livello essenziale delle prestazioni. potrebbe essere astrattamente considerata livello essenziale delle prestazioni. Ma la domanda inevasa è se la legislazione vigente sia o meno adeguata e attuata in maniera uniforme su tutto il territorio; insomma, se sia o meno conforme alla Costituzione. allora non abbiamo atteso che il CLEP terminasse il proprio lavoro e ci mettesse a conoscenza dello stato di attuazione dei diversi livelli essenziali o perlomeno dei criteri che verranno seguiti per la loro determinazione e delle risorse che sarà necessario reperire?

con cui il Governo propone, in maniera peraltro piuttosto pasticciata, di eleggere direttamente il Presidente del Consiglio, di marginalizzare il ruolo e la funzione del Parlamento e con esso del Presidente della Repubblica; in breve, di ridurre la democrazia alla scelta del Capo. Si è consumato uno scambio tra le due riforme, tra la Lega e Fratelli d'Italia - e la prima, sull'autonomia differenziata, ha avuto la meglio uno scambio al ribasso, perché, nel merito, ha prodotto disposizioni del tutto irragionevoli, che rischiano di far crescere divisioni e conflittualità territoriali, politiche e sociali e così, alla fine, di impoverire tutto il Paese. Nei pochi minuti che mi rimangono potrò evidenziarne solo alcune. Ignorando i moniti della Banca d'Italia, dell'Ufficio parlamentare di bilancio e di illustri componenti del Comitato, come Giuliano Amato, Franco Bassanini, Franco Gallo e Alessandro Pajno, il disegno di legge in esame prevede

un'inversione tra articolo 117 e articolo 116 che solleva seri dubbi di costituzionalità. Il Titolo V, pur con tutti i suoi limiti, è chiaro nel prescrivere che si dia prima attuazione all'articolo 117, che prima cioè si attuino i LEP, e solo dopo si possa eventualmente procedere ad attribuire forme di autonomia differenziata ad alcune Regioni. L'articolo 116, terzo comma, non è autoapplicativo e non impone affatto di devolvere competenze legislative, di dividere il Paese o di far crescere disuguaglianze, ma si limita ad ipotizzare un'eventualità, che dovrebbe essere concretizzata con prudenza e nella misura in cui vi siano adeguate condizioni di uguaglianza e produca benefici all'intero Paese. Ancora, nonostante l'articolo 117 della Costituzione sia chiarissimo nel prescrivere che i livelli essenziali vengano determinati con legge o eventualmente con atto avente forza di legge, l'articolo 3 del disegno di legge Calderoli, anche dopo essere stato emendato, continua a prevedere che i livelli essenziali delle prestazioni siano determinati e aggiornati con Forse non avete avuto il tempo di leggere con attenzione la riformulazione proposta dal Governo, ma il comma 9 e poi il comma 10 dell'articolo 3 specificano che, nelle more dell'approvazione dei decreti legislativi, i livelli essenziali continueranno a essere determinati con DPCM e che, alla data di entrata in vigore dei decreti, è fatta salva la determinazione dei LEP avvenuta con DPCM. Per chiudere il cerchio, lo stesso articolo 3 prevede che i LEP potranno essere aggiornati periodicamente, in coerenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con DPCM. Il testo originario è stato emendato, certo; ma, se questi sono i risultati, faccio fatica a capire come i presentatori dell'emendamento, che mi sembra siano i massimi esponenti di Fratelli d'Italia in Commissione, possano esultare. O forse esultano perché, in coerenza con la riforma costituzionale del premierato, si concentra così ogni potere nel Presidente del Consiglio. L'articolo 2, del resto, non chiarisce neppure se le Camere possano emendare le intese o solo pronunciarsi con un sì o con un no e soprattutto non garantisce alcun effettivo ruolo alle Camere nella fase di definizione delle intese. Ci troviamo insomma di fronte a una legge dalla dubbia efficacia giuridica, che marginalizza il ruolo del Parlamento a favore del Governo, e soprattutto che, nel ribaltare il rapporto tra gli articoli 116 e 117 della Costituzione, rischia di accrescere disuguaglianze e divisioni

ricche. Come ci hanno spiegato gli auditi e ci ha ricordato il presidente Mattarella, le profonde disuguaglianze che attraversano il nostro Paese non sono il prezzo che occorre pagare per promuovere crescita e sviluppo, ma, al contrario, una zavorra che pesa su di essi. Per queste ragioni, per non accrescere ulteriormente la zavorra delle disuguaglianze, per preservare l'unità e l'indivisibilità della Repubblica, il nostro voto sarà contrario e la nostra opposizione continuerà ad essere ferma e determinata.

sarò costretto a sospendere la seduta e non vorrei farlo, visto che siamo in diretta TV.

rappresentanti del Governo, colleghi, ci apprestiamo ad approvare in Senato il disegno di legge sull'autonomia differenziata,

*(Applausi)*. In questi giorni, ma anche in precedenza, abbiamo ascoltato dalle opposizioni gli effetti catastrofici che questo provvedimento dovrebbe determinare.

a più livelli, con sanità di serie A, di serie B e forse di serie C, con ampie zone di disagio, con trasporti che funzionano molto bene in alcune Regioni e infrastrutture che in altre non ci sono proprio;

e che, giorno dopo giorno, stiamo aiutando a rimettersi in piedi, con il nostro impegno. *(Applausi)*. Altro che spacca Italia! Il Governo l'Italia la sta ricucendo, anche e soprattutto portando nelle zone disagiate e svantaggiate piani di investimento che aiutino la crescita e superino l'abbandono che c'è stato per anni, oppure l'assistenzialismo tossico del reddito di cittadinanza. Con il provvedimento in esame diamo attuazione a una norma che per anni è rimasta nel cassetto, ovvero impegniamo il Governo e il Parlamento a individuare i livelli essenziali delle prestazioni prestazioni legati alle materie che impattano sulla vita dei cittadini che - per usare le autorevolissime parole del professor Cassese - mettono il fuoco sotto la sedia al decisore pubblico, che, nel momento in cui vengono determinati i livelli essenziali delle prestazioni,

con una serie di informazioni che possiamo serenamente definire propagandistiche e lontanissime dalla realtà del testo che ci accingiamo ad approvare;

categoricamente escluso, a maggior ragione dopo il lungo lavoro svolto in particolar modo in 1a Commissione. Devo ringraziare per la sapiente regia di questo lavoro il presidente Balboni

sul tema della coesione e dell'unità nazionale inserito nell'articolo 1, quindi già nei principi di base del provvedimento, e quelli relativi al fatto che si debbano fare decreti legislativi, quindi che ci sia il controllo del Parlamento nei provvedimenti di determinazione dei LEP.

gli altri emendamenti su cui hanno fatto un grande lavoro i parlamentari di Fratelli d'Italia delle isole e del Mezzogiorno - che ci hanno messo la faccia e non hanno certo paura di affrontare inesistenti critiche - che hanno inserito i temi dell'insularità e del *gap* infrastrutturale all'interno dei livelli essenziali delle prestazioni; l'emendamento approvato dall'Assemblea che garantisce in modo inequivocabile che i presunti svantaggi non ci saranno. Quest'ultimo punto si può spiegare in un modo molto semplice: se la richiesta di una materia da parte di una Regione che vorrà chiederla, in relazione a quanto previsto dall'articolo 116 della Costituzione, dovesse costare un euro in più come spesa generale, quell'euro in più dovrà essere speso anche per le Regioni che l'autonomia non la chiederanno. Non ci sarà quindi alcun danno per le Regioni che non chiederanno l'autonomia. *(Applausi)*. L'autonomia differenziata è solo un'opportunità e siamo convinti che la potranno cogliere, contrariamente a quello che viene raccontato, anche le Regioni

e questo ci fa dire che tale intervento può stare perfettamente e a pieno titolo nel percorso delle riforme che stanno già procedendo, come quella del premierato, e di quelle che verranno realizzate. A questo proposito, è importante anche che l'Assemblea abbia accolto un ordine del giorno che fa riprendere quel percorso, mai portato a compimento, per dare poteri e risorse adeguate anche alla Capitale d'Italia, come avviene in tutti i principali Paesi europei e non solo. *(Applausi)*. E si farà la riforma della giustizia. colleghi, è accaduto spesso nella storia, non solo italiana, ma anche delle grandi democrazie, che i progressisti abbiano parlato in modo inconcludente di riforme e poi alla fine siano diventati i difensori dello *status quo*, mentre i conservatori, che vogliono conservare i valori e le tradizioni, siano stati proprio coloro che hanno fatto le riforme per modernizzare lo Stato. È accaduto, sta accadendo e accadrà in questa legislatura. Presidente, qualcuno anche nella discussione odierna ha parlato di baratto. Giorgia Meloni, il suo Governo, Fratelli d'Italia e il centrodestra non avrebbero mai messo nel programma, che è stato unitario - come altri hanno ricordato - qualcosa in cui non si crede e qualcosa che possa essere dannoso per l'Italia. Noi potremmo anche sbagliare, non siamo perfetti, ma siamo qui per servire l'Italia non abbiamo alcun baratto da fare; non so se lo stesso possano dire altre forze politiche. Sono rimasto un po' stupito durante la discussione qualche giorno fa quando il Gruppo MoVimento 5 Stelle, di solito molto agitato quando c'è una discussione, è rimasto impietrito - sembravano statue di sale - quando il ministro Calderoli ha ricordato il contratto di Governo che prevedeva

più vicino ai cittadini attraverso le Regioni e ancor meglio attraverso i Comuni, le Province e le Città metropolitane, e anche questo è contenuto nel testo in esame. Soprattutto però non si spacca e non si divide nulla,

borghi e delle differenze enogastronomiche. Quell'Italia delle tradizioni popolari e religiose, però, dalla più piccola frazione alla più grande metropoli, ha luoghi che simboleggiano la sua unità, cioè i monumenti ai caduti. è fisicamente visibile come si sia forgiato, nel sacrificio delle trincee, quel sentimento nazionale che per noi è sacro e non è minimamente intaccato da questo provvedimento, al quale, sapendo di aver fatto un buon lavoro, a testa alta dichiariamo il voto favorevole di Fratelli d'Italia.

il collega Lombardo il fatto che, se verrà approvato, il banco di prova per il Governo rimarrà il finanziamento di tutti i diritti di cittadinanza e dei servizi che devono essere garantiti a tutti i cittadini, come prevede la Costituzione. Resta però il fatto che l'impianto regolatorio del provvedimento mi convince per tre ragioni: innanzitutto, perché me ne ero occupata durante il Governo Draghi e penso che non si debba cambiare idea solo perché si passa dalla maggioranza all'opposizione. nel provvedimento in esame ci siano due punti. Il primo è che si archiviano le intese dirette tra le Regioni e lo Stato e si preferisce una legge quadro, una legge cornice, che giustamente è stata pensata anche per rappresentare le istanze e i diritti delle Regioni che decidono di non accedere a un percorso di autonomia, ma che devono vedere garantite le loro prerogative. Non solo: durante il Governo Draghi mi ero battuta per il finanziamento dei diritti di cittadinanza, per la definizione di tutti i diritti di cittadinanza, ed è indubitabile che il finanziamento un percorso che non comincia oggi, ma la definizione, grazie al lavoro del professor Cassese, è stata fatta. Penso che l'aspetto più importante del provvedimento sia il passaggio dalla spesa storica,

le classi dirigenti si dovranno confrontare, ma non dovranno farlo per chiedere più risorse, bensì si dovranno soffermare su come vengono spese le risorse. E sono certa che in quell'ambito vi sia la possibilità di un grande efficientamento della spesa pubblica e per un Paese fortemente indebitato come l'Italia questo è un punto importante. Concludo dicendo che, indipendentemente da come la si pensi sull'autonomia, la definizione e i finanziamenti dei LEP, cioè il passaggio dalla spesa storica al costo *standard* e al fabbisogno *standard*, saranno un elemento centrale all'interno della riforma del federalismo prevista tra le riforme fondamentali del PNRR e alla quale è legata una *tranche* di 32,8 miliardi dentro il PNRR. Per tutte queste ragioni, confermo il voto a favore del provvedimento.

Colleghi, sospendo la seduta.

Colleghi, sentiti i Capigruppo, anche in relazione ad alcune riunioni di Gruppo, concludiamo ora

Presidente, colleghe e colleghi, nella serata di ieri il cuore grande di Gigi Riva si è fermato. *(Applausi)*. Cagliari e tutta la Sardegna sono in lutto. La solidarietà, l'affetto e il dolore di milioni di italiani sono nelle parole che ieri il presidente della Repubblica Mattarella ha dedicato alla memoria di questo campione, di quest'uomo immenso. Sfuggire alla retorica e alla commozione nel ricordare Gigi Riva per le generazioni di sardi, tra le quali la mia, cresciute nel suo mito, è davvero difficile. Nato a Leggiuno, in provincia di Varese, nel 1944, Riva giunse in Sardegna nel 1963, quando la nostra Regione era un luogo nel quale venivano mandati i militari e i funzionari pubblici come punizione, più che il meraviglioso luogo di villeggiatura, noto in tutto alla fine di quel decennio per molti italiani. Riva ci arrivò dopo un'infanzia di privazioni materiali; era nato in una famiglia molto povera e di dolore autentico per la perdita in giovanissima età di entrambi i genitori. Arrivò ragazzo, si fece rapidamente uomo e rimase in Sardegna per tutta la carriera e poi per tutta la vita, resistendo a lusinghe di successi e di denaro apparentemente irresistibili. Se non si comprende la durezza della condizione della Sardegna di quegli anni, nei quali ricominciavano a essere concepite le infrastrutture della rinascita nel tentativo di sottrarla all'arretratezza; se non si conosce la condizione dei nostri immigrati costretti dalla povertà estrema a raggiungere la Svizzera, la Germania e il Nord Italia per svolgervi i lavori più umili, in condizioni ora inimmaginabili; se non si ricorda un'altra piaga della Sardegna dell'epoca, il banditismo e i sequestri di persona, e se non si ricorda quale fosse anche per queste ragioni la considerazione della Sardegna nel resto d'Italia e di noi sardi nei confronti di noi stessi; se non si conoscono tutte queste cose, non si può capire cosa sia stato per la Sardegna Gigi Riva e il significato dell'epopea di una squadra di calcio che riscatta un'intera Regione e fa percepire a tutto un popolo di potersi misurare, vincendo, con tutta l'Italia, compresa quella più ricca. riconobbe di essersi fatto sardo, di aver scelto di essere sardo. Quando gli chiesero come mai, disse che succedeva a tutti quelli della squadra di allora, perché quando fuori li chiamavano pecorari e banditi, era inevitabile che si "incavolassero" e allora vincevano di più. «sicuramente i torti che subivamo allora noi sardi hanno contribuito a farmi identificare con questo popolo. Ma insieme ai valori che ho incontrato. Sono cinquanta anni che giro l'Isola, sono di casa ad Orgosolo, Mamoiada. Ho incontrato gente meravigliosa». Ecco, lui ha deciso di diventare sardo, è stato sardo per scelta. Riva è stato però anche un grande italiano, è stato uno degli eroi nazionali della Sardegna del Novecento, insieme forse solo ad Emilio Lussu. Lui che amava la Sardegna visceralmente e ha legato per sempre la sua vita alla sua e nostra amatissima bandiera del Cagliari, sentiva l'appartenenza alla nazionale italiana di calcio come un onore assoluto, il più alto, e oggi la sua salma è stata composta con la tuta azzurra della nazionale che vestiva in quegli anni. Con la nazionale ha avuto grandissimi successi e amare sconfitte, prima da calciatore e poi da *team manager*, per finire con la vittoria mondiale a Berlino nel 2006. Rimane da decenni il calciatore più prolifico di tutti i tempi in maglia azzurra. Gigi Riva con la sua coerenza, il suo rigore e la sua serietà è stato un grande sardo e un grande italiano. In nel descrivere il dolore e l'angoscia per il drammatico infortunio occorso a Riva con la maglia della nazionale il 31 ottobre del 1970, Gianni Brera scrisse: «Io vorrei solo che degli eroi autentici non si guastasse mai il ricordo. L'uomo Riva è un serio esempio per tutti. Il giocatore chiamato Rombo di tuono» - così lo aveva chiamato lui, per quasi incredulo entusiasmo - «è stato rapito in cielo, come tocca agli eroi». Ora quel destino è toccato all'uomo che tanto abbiamo amato. Certamente non si guasteranno mai il suo ricordo e il suo esempio.